di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

In effetti, non si tratta di un riconoscimento per meriti speciali, ma si tratta di disciplinare i percorsi formativi e la definizione dei profili delle prestazioni che vengono erogate dai dottori in scienze delle attività motorie e sportive a garanzia primaria della salute pubblica. Credo che sia questa l'occasione per colmare un vuoto normativo e per fare un passo in avanti affinché i profili di garanzia che derivano dalle norme che disciplinano la regolamentazione delle prestazioni professionali possano andare nella direzione di riconoscere senz'altro un'attività notoriamente ormai consolidata nell'ambito del panorama sanitario, ma anche nella direzione primaria

e ha, tra gli appuntamenti di rilievo, la giornata di formazione per i medici di medicina generale della Romagna, che tratteranno della prescrizione dell'esercizio fisico in ricetta medica per la prevenzione e la terapia delle principali malattie croniche. Ritengo che questa sia un'ulteriore manifestazione di quanto sia importante l'esercizio fisico ben fatto come prevenzione delle patologie e delle malattie. Questo è ormai scientificamente provato, quindi il fatto che questo emendamento sia stato trasformato in un ordine del giorno mi fa sperare che finalmente si continui a ragionare di questo e non cada tutto nell'oblio per altri vent'anni.

alle ore 16,54)*. Invito i colleghi a prendere posto dovendosi procedere a votazione elettronica.

in sede di recepimento di direttive comunitarie, ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali,

che rimanga agli atti che noi istituiamo la figura professionale dell'osteopata, non secondo le richieste del senatore Volpi, ma con un emendamento, diventato testo, votato in Commissione. Un emendamento importante, che ha visto la convergenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute. Si istituisce una professione attraverso la definizione di un percorso di laurea triennale, con il mandato ai Ministeri a definire, in sede di attuazione, i profili formativi e professionali. Lo dico, signor Presidente, perché c'è stata molta polemica su questo argomento. Ritengo sia un passo importante. Noi validiamo ciò che già c'è nella società, dando però garanzie e uniformità di formazione

ci sono contenziosi aperti per uniformare la formazione del medico specialista alle direttive europee. Con questo emendamento si dice in realtà di di rispettare i criteri europei e di valutare la qualità della formazione, affinché non sia fittizia ma di fatto.

n. 368, e successive modificazioni». Il comma in oggetto dispone che possano essere definite ulteriori modalità di attuazione per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno del Sistema sanitario nazionale. Con questa norma c'è la forte preoccupazione che, non risolvendo affatto la criticità della formazione specialistica, si avalli l'utilizzo degli specializzandi per supplire alle carenze di organico del Sistema sanitario nazionale, creando così un ulteriore ostacolo all'accesso al mondo del lavoro per i medici neospecialisti. Supplire quindi alle gravi carenze di organico del Sistema sanitario nazionale attraverso i medici in formazione specialistica, che di fatto andrebbero a svolgere mansioni assumendosi responsabilità proprie del personale strutturato, è in palese contrasto con il principio di non sostituibilità del personale di ruolo, sancito dall'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999. 10.201 dispone: «Il rapporto tra medici in formazione specialistica e personale strutturato dirigente medico non può essere inferiore al rapporto di uno a sette»

4. Abbiamo discusso in Commissione, trovando un consenso molto ampio, di un argomento di straordinaria importanza: la formazione specialistica dei medici e la relazione fra la formazione universitaria e le Regioni. Speravamo che la contrarietà originaria della Commissione bilancio potesse nel frattempo attenuarsi e trasformarsi in un parere favorevole.

ricerca. È lo stesso ragionamento che porta, nella discussione sull'articolo 22 del cosiddetto Patto per la salute, una certa stasi nel dibattito,

venga ripreso dal Patto per la salute, perché non possiamo continuare a pensare che i nostri medici possano vedere una persona in carne ed ossa, malata, un paziente, dopo 30 anni. Francamente siamo fuori dal mondo! [DE relatrice e confermo l'impegno del Governo a procedere speditamente sull'articolo 22 del Patto per la salute, che dovrebbe chiarire una materia non semplice, ma sulla quale stiamo lavorando operosamente, come sa la presidente

lettere indirizzate alla Camera dei deputati e allora vorrei recuperare le ragioni, che in modo puntuale e preciso, sono state esposte nella scorsa seduta dal collega senatore Zizza in ordine

in relazione a un capitolo particolarmente importante, rimasto irrisolto nella precedente legislatura e che non vorremmo rimanesse irrisolto in questa.

distintivo che deve mettersi una categoria che si costituisce in ordine, ma per i progressi tecnico-scientifici che nell'ambito dell'ottica e dell'optometria sono stati conseguiti. Tali ragioni inducono a disciplinare in modo puntuale e preciso i requisiti formativi, anche per evitare che prolifichino o proliferino le scuole di formazione, che fanno *business* attorno a questi percorsi formativi senza i necessari livelli di validazione, che invece meritano di essere ben disciplinati e puntualmente riconosciuti, al fine di un maggiore livello di tutela della salute dei cittadini.

Commissione. **È approvata.** Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio S.100, riferita all'articolo 9 e agli articoli da 11 a 25 del testo originario del disegno di legge, le disposizioni ivi contenute confluiranno in un autonomo disegno di legge, che sarà immediatamente deferito alle competenti Commissioni parlamentari.

di legge che riformula la sperimentazione clinica delle fasi da zero

questa insistenza, perché abbiamo la possibilità, anche per quanto riguarda l'archivio informatizzato, di avere l'albo nazionale per ogni

di 6.000 in Italia, quasi quanti negli Stati Uniti - dobbiamo considerare che quello che abbiamo in Italia e che chiamiamo osteopata non è la stessa figura dell'osteopata che esercita negli Stati Uniti: lì gli osteopati sono medici specializzati, hanno tutto un altro profilo, hanno almeno sette anni di studi. Gli osteopati che abbiamo in Italia, spesso, sono persone che hanno fatto corsi a pagamento, che hanno fattoil *business* di molti, nel *weekend*, per un periodo limitato e non sono neanche medici.

del genere, sia un'incongruenza, mentre altre figure, molto più definite, avrebbero meritato più attenzione. Non si capisce perché qualcuno sì e qualcuno no. Poi mi dovete spiegare la differenza: perché l'osteopata sì e il chiropratico no?

questo fa sì che vi sia la solita incongruenza normativa, una non armonizzazione della legge, che genererà confusione. Ma ho un ulteriore motivo di riserva: diamo la disponibilità

immettiamo nuove figure che devono essere formate, ma a discapito di chi? Come facciamo a rientrare nei numeri, nei costi? Riduciamo la formazione, portando la scuola di specializzazione da cinque a quattro anni e magari

abbia confermato come e quanto, sia pure nella differente sensibilità politica, grazie ad un lavoro orientato verso la qualità di una produzione legislativa adeguata alle aspettative del Paese, possa consegnare al Paese stesso un prodotto legislativo adeguato ai tempi. Devo dire preliminarmente che il voto

figlio di quello che nella scorsa legislatura fu l'Atto Camera 4274, approvato dalla Camera dei deputati con il Governo di centrodestra, giunto con quel Governo in quest'Aula in quest'Aula con l'Atto Senato 2935 e purtroppo non arrivato alla sua definitiva approvazione per le questioni politiche che portarono alla caduta di quell'Esecutivo. Ebbene, io voglio esprimere al ministro Lorenzin e al sottosegretario De Filippo l'apprezzamento, perché di quel disegno di legge hanno recuperato i tre quinti;

la Commissione sanità ha approfondito in modo puntuale e preciso i suoi contenuti con un dibattito che è stato di qualità. Lo stesso dibattito è

anche da posizioni politiche diverse, con sfumature differenti, ha portato alla fine ad esprimere una valutazione positiva. Credo che questo, Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, sia un buon modo di lavorare, e mi permetto di sottolineare, in questo modo anche recuperando un doveroso pensiero di

il livello del nostro impegno anche in Assemblea. In discussione generale ho già esposto le mie osservazioni su questo le sintetizzo facendo un volo rapido sugli aspetti di maggior rilievo, quelli all'articolo 1, sulla sperimentazione clinica dei medicinali, che tiene conto del processo necessario di armonizzazione della legislazione domestica rispetto a quanto accade in Europa, ma afferma in piena autonomia i princìpi di maggiore trasparenza, di terzietà, di indipendenza della ricerca scientifica. Si recupera quindi un aspetto importante, quello della medicina di genere che, come ha detto la collega relatrice, non è l'aspirina rosa, ma è in effetti il progresso delle scienze farmaceutiche, che allunga lo sguardo ieri ai problemi dell'età pediatrica, avant'ieri a quelli del diverso metabolismo dell'anziano, oggi alla medicina di genere, traguardando evidentemente

Dopo settant'anni si riconosce agli organi professionali la loro funzione pubblicistica, il loro *status* giuridico di enti di diritto pubblico sussidiari dello Stato. In quell'aggettivo credo credo ci sia tutta la valenza, la forza di un ente pubblico che territorialmente è destinato non a far rivivere in modo improprio residui di corporativismo che fanno male alle professioni, ma a rilanciare le funzioni di natura pubblicistica a beneficio della comunità. Ricordo ancora l'aspetto relativo all'esercizio abusivo delle professioni: peraltro, questo è un tema che è stato ampiamente dibattuto in Senato con l'approvazione di un disegno di legge che oggi, con l'Atto Camera 2281, è all'esame dell'altro ramo del Parlamento. la farmacia dei servizi: credo che l'articolo 11, con la previsione della legittimazione all'esercizio delle professioni o delle arti sanitarie all'interno della farmacia - con l'ovvia esclusione, nel rispetto nel rispetto dell'antica ma ancora moderna volontà del *puer Apuliae*, mantenendo dunque la separazione tra l'atto prescrittivo e l'atto dispensativo - indubbiamente consente di attuare la famosa legge n. 69 del 2009, che vuole rilanciare la funzione della farmacia come presidio sociosanitario del territorio rappresentando un punto di primo approccio della comunità rispetto ai problemi della salute. Si poteva fare di più? Sì, si poteva fare di più. Però sappiamo che il meglio è nemico del bene. Potevamo fare di più sulle questioni inerenti le aspirazioni di alcuni ordini professionali, ma credo che i messaggi inviati alla Camera dei deputati attraverso l'approvazione di ordini del giorno la dicano lunga sulla sensibilità. sensibilità. Per quanto riguarda il mio Gruppo, credo che il senatore Zizza abbia espresso in modo puntuale e preciso quanto riconfermo adesso in relazione all'auspicio e alla necessità

Credo che alla Camera dei deputati questi problemi verranno affrontati. Per quanto riguarda la formazione specialistica, la relatrice, con grande onestà intellettuale, ha detto che volevamo anche noi fare qualcosa in più. qualcosa in più. Relativamente all'articolo 22 del Patto della salute volevamo fare un passo in avanti, ma naturalmente le incomprensioni e i conflitti, per alcuni versi, tra il MIUR e il Ministero della salute, hanno visto tirare il freno a mano su un argomento che resta centrale nell'ambito del dibattito che, sono convinto, verrà affrontato e risolto in sede di esame nell'altro ramo del Parlamento. Concludo sull'ultimo punto dei farmaci innovativi. Se vogliamo realmente dare un segnale di serio investimento sulle farmacie come presidio sociosanitario del territorio, dobbiamo riportare i farmaci innovativi all'interno della farmacia per una dispensazione che costi di meno e giovi di più sotto il profilo del controllo e del monitoraggio dei consumi, naturalmente fatti salvi quei farmaci la cui somministrazione necessita obbligatoriamente di un monitoraggio in sede ospedaliera. Credo che questo significhi andare in una direzione di efficientamento complessivo delle terapie, ma anche di un miglior governo della spesa. Credo che recuperare i farmaci innovativi nelle farmacie voglia dire non soltanto

quella potestà prescrittiva e dispensativa che oggi non esiste, cosa che ha determinato un vero impoverimento di queste due professioni. Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Conservatori e Riformisti, formulando l'auspicio che i punti di criticità, che ho esposto, possano essere recuperati in un dibattito che, sono convinto, alla Camera

il testo approvato con voto unanime in Commissione è piuttosto articolato e tratta una pluralità di tematiche alquanto differenziate. Tra i temi di maggiore rilievo si segnalano le disposizioni concernenti il riordino delle professioni sanitarie, che sono state valutate sia alla luce degli indirizzi politici promananti dall'Unione europea, sia in considerazione della necessità di disciplinare in maniera omogenea le diverse professioni, così da riconoscerne la pari dignità e da valorizzarne le competenze, necessarie alla funzionalità del sistema sanitario. In questo provvedimento vengono poste le premesse perché siano finalmente date risposte a istanze di adeguamento dell'ordinamento pendenti da decenni, dalla revisione della disciplina delle sperimentazioni cliniche fino a quello che rappresenta il cuore del provvedimento, ossia il riassetto della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie e la regolamentazione di alcune professioni sanitarie che vengono, allo stato, esercitate in assenza di una cornice normativa. In particolare, per quanto attiene al riordino delle professioni sanitarie già disciplinate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, si auspica che con l'entrata in vigore della nuova normativa gli ordini potranno svolgere più efficacemente le proprie funzioni, che in ultima analisi sono volte a garantire un adeguato livello qualitativo alle prestazioni sanitarie rese agli utenti. Con l'intervento operato si sostituisce gran parte del predetto decreto legislativo n. 233 del 1946, e le nuove norme organizzative concernono sia gli ordini esistenti dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sia i nuovi ordini summenzionati. Si trasformano gli attuali collegi delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali accorpando in un medesimo Ordine, quello dei tecnici sanitari di radiologia medica, professioni tra loro omogenee e compatibili, quali le professioni sanitarie tecniche della prevenzione e della riabilitazione che pur regolamentate non hanno ancora albi professionali. Appare importante ricordare come osteopati e chiropratici diventano professioni sanitarie. Tra le principali novità del testo approvato dalla Commissione figura senz'altro l'istituzione di due nuove figure professionali, quella dell'osteopata e del chiropratico, che diventano a tutti gli effetti professioni sanitarie. Gli osteopati avranno anche un apposito albo all'interno del neo-Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Una criticità che non è stata risolta è quella relativa al riconoscimento dei titoli con i quali l'osteopata viene definito come il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente, svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione europea degli osteopati e dall'Organizzazione mondiale della sanità secondo criteri funzionali relativi alla prevenzione della salute dell'individuo. Ci si augura che l'errore venga corretto attraverso il compimento di quanto previsto dall'articolo 4, inserito in sede referente, dove per l'iscrizione è richiesto il possesso della laurea abilitante in base all'ordinamento didattico da definire secondo la procedura di cui al comma 2 del presente articolo 4 - o dei titoli equipollenti -individuati con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

per la verità con enorme ritardo, è un provvedimento che avrebbe dovuto già essere stato perfezionato e promulgato da sei anni. Ricordo a me stesso e agli astanti che tale disposizione,

non vide poi la luce perché, nel successivo passaggio al Senato, incontrò la fine anticipata della legislatura. Questo può essere anche portato ad esempio dell'opportunità per quest'Assemblea e per l'altro ramo del Parlamento di aver licenziato il progetto di riforma costituzionale,

Partiamo dall'elemento più importante, vale a dire la disciplina ovvero il percorso giuridico scientifico riguardante la sperimentazione clinica. Noi siamo un Paese nel quale, ricorrentemente, dal siero anticancro del professor Vieri (che altro non era che colchicina, quindi un inibitore della mitosi nucleare) al siero di Bonifacio, alla cura Di Bella, alla cosiddetta cura Stamina, ogni tanto troviamo qualcuno che ventila la scoperta di una cura per la malattia del secolo,

all'insistenza dei familiari e dei malati, ha sempre decretato la sperimentazione di ciò che pareva essere il rimedio o la cura di questa malattia, sessant'anni non ci siamo mai muniti di un provvedimento legislativo che indicasse un percorso scientifico e giuridico a cui andava - andrà - avviata ogni ipotesi sperimentale sia per i farmaci che per le cure.

delle nanotecnologie, delle cure che si attagliano all'individuo e non alla malattia della sperimentazione avanzata sia tecnologica che immunologica per fronteggiare malattie ancora resistenti alle cure.

che hanno la necessità di essere riconosciuti nell'ambito delle attività e delle professioni sanitarie. Mi piace ricordare i biologi, la cui legge istitutiva risale al 1967, per tutta una serie di ritardi, non sono mai stati riconosciuti come categoria sanitaria. L'Ordine era sotto l'egida addirittura del Ministero di grazia e giustizia, la qual cosa era veramente fuori da ogni logica e ogni criterio e - soprattutto - senza la possibilità di un continuo e costante controllo sulle attività degli ordinisti.

che qualcuno continua a ritenere non degne di un titolo scientifico - ma io non sono tra questi - siano puntualmente identificati. Questi professionisti,

in grado di poter essere equiparato a quello di tutte le altre professioni sanitarie che, com'è noto, necessitano non solo della laurea magistrale ma anche di una puntuale specializzazione per poter accedere

mettere sul mercato professionisti che non hanno un bagaglio culturale e una preparazione tali da poter essere sovrapponibili al percorso di studi e di preparazione delle altre categorie.

che quando parla di sanità pubblica o di servizio pubblico non deve commettere l'errore di confonderli con il servizio statale. Anche le farmacie private, persino i bar o i ristoranti si chiamano servizi pubblici. La si smetta, una volta per tutte, di confondere la pubblicità con la statalità. Lo Stato non persegue etiche superiori; l'unica etica in sanità è l'interesse e la cura del malato, e l'unico interesse dello Stato è accertare la qualità della cura la compatibilità dei costi alle disponibilità. Il resto è aria fritta. Il resto è mantenere, all'interno di un comparto, quei privilegi di cui godono gli statali, che millantano di avere un'etica superiore dei fini, ma in realtà producono puntualmente disavanzi e disservizi con liste d'attesa che nel comparto non statale non esistono. Questa

del presidio o del professionista. Mi auguro che in quest'Assemblea il concetto che vado ripetendo da tempo possa diventare patrimonio di tutti coloro i quali hanno a cuore il Sistema sanitario e soprattutto i malati. Salutiamo studentesse e studenti dell'Istituto tecnico e tecnologico statale «Fedi-Fermi» di Pistoia. Benvenute e benvenuti al Senato.

la delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e riordino delle professioni sanitarie ha finalmente concluso il suo *iter* legislativo nel Senato della Repubblica. Dico anch'io «finalmente» perché questo disegno di legge si occupa di aspetti molto rilevanti in riferimento alla tutela della salute pubblica, sia in termini di miglioramento della sicurezza delle cure erogate ai cittadini, sia nel senso di una migliore organizzazione delle professioni sanitarie, contribuendo così ad una generale crescita di qualità del nostro sistema sanitario. Gli interventi in discussione generale e quelli che oggi mi hanno preceduto hanno già ben sottolineato gli aspetti innovativi, peraltro attesi da anni, di questo provvedimento. Vorrei soffermarmi anche io su alcuni punti, che ritengo meritevoli di sottolineatura. Il primo è contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge e riguarda il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazioni cliniche. io: era ora! Ricordo che proprio all'inizio di questa legislatura, prima ancora che ci fosse la nomina delle Commissioni permanenti, ci dovemmo occupare di quel caso paradossale e drammatico, chiamato poi caso Stamina, false illusioni vendute a tante famiglie disperate e professionalità mediche compromesse e rese ridicole da inspiegabili comportamenti professionali. Mi auguro che questa brutta vicenda, tutta italiana - ci è stato ricordato che non è la prima - possa essere soltanto un lontano ricordo e che il Governo, con questa delega forte del Parlamento, possa finalmente definire con precisione

dall'individuazione dei centri autorizzati, alle adeguate sanzioni per chi si permette di truffare i cittadini. la guida migliore nell'operare deve essere la coscienza onesta e limpida. Non mi soffermo sui nuovi LEA, che riguardano le procedure di controllo del dolore nel parto, già mirabilmente illustrati dal collega senatore Lucio Romano. Alcune considerazioni le merita il riordino della disciplina

delle professioni infermieristiche, di ostetrica, dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e prevenzione, nonché dell'Ordine dei biologi e degli psicologi, oltre alle nuove norme organizzative per gli ordini già esistenti dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti, hanno come scopo quello di organizzare al meglio la sanità, mettendo i professionisti di questo settore strategico nelle migliori condizioni per per operare ed esprimere al meglio la propria professionalità. Una considerazione personale riguarda le due nuove professioni che il disegno di legge in esame si propone di istituire: l'osteopata e il chiropratico. Abbiamo sentito tante considerazioni la scelta del provvedimento è stata di proporre due nuove professioni, ma un'alternativa sarebbe potuta essere quella di inserirle nel percorso di studio di professioni sanitarie che già da tempo fanno uso di tecniche della medicina manipolativa manuale,

che si creassero in futuro equivoci o malintesi che avrebbe ricadute negative inevitabili sugli cittadini. Comunque la via è stata presa e, concluso il passaggio parlamentare, mi auguro che i passaggi governativi e i chiarimenti tecnici necessari possano arrivare a fare ordine nel settore importante della riabilitazione, comprese quindi anche queste due nuove discipline. Un ulteriore aspetto molto positivo è dato dalla volontà di riorganizzare il percorso formativo degli specializzandi in medicina. Ci sono ancora molti punti critici nella formazione dei futuri specialisti. Ad esempio, spesso ci sono più opportunità formative nei piccoli ospedali periferici che in blasonate cliniche universitarie e questo è un segnale che qualcosa non funziona. Prima di concludere, vorrei ringraziare di cuore la presidente della 12a Commissione, Emilia De Biasi, per la tenacia

È vero, come ha detto il senatore D'Ambrosio Lettieri, che il meglio è nemico del bene, ma penso che in una discussione seria e approfondita approfondita far capire perché su alcuni punti dobbiamo cercare sempre il meglio è importante, anche se poi dobbiamo accontentarci del risultato finale. Sicuramente in Commissione sanità abbiamo fatto un ottimo lavoro: abbiamo portato avanti il tema della medicina dei servizi e abbiamo riorganizzato tutto il concetto degli ordini dei medici, anche se come ho detto in discussione generale - avrei sicuramente preferito che, all'interno degli ordini dei medici, ci fosse stata una maggiore democrazia, permettendo anche alla lista che perde di avere una sua rappresentanza. Questo forse è un sogno, ma prima o poi spero si realizzi, per portare più professionisti a votare per il proprio ordine dei medici, vista la scarsa affluenza. Devo spezzare Devo spezzare una lancia anche a favore dei chiropratici e degli osteopati. Sono perfettamente convinto che queste siano due figure utili in ambito sanitario, che da molto tempo collaborano con molti medici,

a spiegare a molti di noi che il grande sforzo che la nostra sanità sta facendo è rivolto principalmente a coloro che sono già malati e, quindi, necessitando delle cure appropriate, risulta molto difficile ridurre l'impegno di spesa. Poiché stiamo andando verso una popolazione sempre più anziana con polipatologie, il fatto che cerchiamo di fare tagli, anzi facciamo tagli di spesa, cerchiamo di seguire il criterio

prevenzione. Credo infatti che sia il modo più efficace per ridurre e razionalizzare la spesa sanitaria. È vero, bisogna cercare di ammalarsi di meno, questa non è un'utopia. Abbiamo visto che seguendo alcune regole

Per cinque patologie è stata approvata la relazione fra l'attività fisica e i benefici sulla salute: parlo delle malattie cardiovascolari, dell'ictus, dei tumori del colon, dei tumori del seno e del diabete di tipo 2. È stato calcolato che, aumentando soltanto dell'1 per cento il numero delle persone attive, si risparmierebbero 80 milioni di euro l'anno di spesa sanitaria. È questo il concetto che voglio far La principale conseguenza dell'inattività fisica è il sovrappeso e la successiva obesità. In Italia il 33 per cento della popolazione è in sovrappeso e il 9,7 è obesa. Come si è arrivati a tutto questo? La medicina scolastica e la medicina militare sono state praticamente smantellate con seria compromissione della prevenzione. L'attività sportiva è importante per la prevenzione di molte patologie e per migliorare le condizioni dei soggetti malati; *exercise is medicine* è il nuovo indirizzo per la prevenzione e la terapia. I ragazzi, inoltre, traggono beneficio dall'attività sportiva anche per la loro maturazione psichica. L'ideale sarebbe istituire nella scuola un corso di educazione sanitaria, nutrizionale e sportiva, al fine di migliorare gli stili di vita e ridurre la spesa sanitaria attraverso l'educazione alla salute, alla salute, alla corretta alimentazione ed alle attività sportive. Bisogna avviare una formazione globale dei docenti della scuola, dei medici di famiglia, degli addetti alla preparazione fisica e atletica e anche dei dirigenti sportivi, perché sono necessari *manager* delle strutture sportive che non siano spinti solo dall'ottenimento del risultato, ma che facciano dell'attività sportiva un mezzo per il miglioramento della salute pubblica. Ma se gli alunni non vogliono fare attività fisica? Nessun problema: li si porta ugualmente sui campi affinché assistano all'attività fisica degli altri e prima o poi - ve lo posso garantire, come è successo a me diventeranno persone che non possono smettere di fare movimento. Questo volevo dire. Per il resto, posso aggiungere che sono d'accordo

però ha anche offerto la possibilità in Commissione di formulare proposte e risposte articolate, che hanno visto protagonisti tutti i Gruppi parlamentari. è già abbondantemente disquisito sul fatto che si tratta di un provvedimento atteso da decenni, che affronta questioni rilevanti dell'organizzazione sanitaria, offrendo risposte puntuali e largamente condivise. A tal proposito, voglio qui ringraziare la relatrice del provvedimento, la senatrice De Biasi, presidente della Commissione sanità, per l'ottimo e appassionato lavoro svolto, nonché i senatori della Commissione sanità, i quali hanno votato il testo all'unanimità dei presenti, a conferma di un lavoro puntuale, unitario ed altamente produttivo. Ad un certo punto del dibattito, in Commissione ci si è resi conto che il testo era troppo esteso, a tratti confuso, in quanto caratterizzato da una eterogeneità di questioni che andavano meglio argomentate ed approfondite. Per questo alcuni articoli sono stati stralciati ed altri sono stati

ricordo la disciplina delle sperimentazioni cliniche, il riassetto della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie e la regolamentazione di alcune professioni sanitarie che oggi vengono esercitate in assenza di una cornice normativa. Il provvedimento contiene anche norme a tutela della professionalità di migliaia e migliaia di lavoratori e della salute di tutti i cittadini. Anche qui, amo ricordare che vengono inasprite le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione, nel caso venga esercitata proprio nel settore in Vorrei altresì ricordare la norma che agevola l'accesso dei giovani alla professione medica. A proposito dei dati sul numero di medici del Servizio sanitario nazionale che andranno in pensione nei prossimi cinque anni, vorrei

medici. Crediamo infatti che sia inaccettabile ed inammissibile che, soprattutto in alcune specialità, vi siano medici che devono garantire prestazioni di qualità trovandosi però in età avanzata, con rischi soprattutto per il cittadino utente. coloro che andranno in pensione nei prossimi cinque anni e sui laureati in medicina ogni anno inducono i vari Ministeri a prevedere una carenza dell'offerta di tale lavoro, professionalmente qualificato, rispetto alla domanda che proviene dalle pubbliche amministrazioni.

proposito ringraziare il Ministero, perché ha dilatato i decreti per quanto riguarda l'accesso alle specializzazioni, portando i posti quasi a 7.000, ma ancora oggi purtroppo ci sono, potenzialmente, 3.000 laureati in medicina che non riusciranno ad accedere alla specializzazione.

sempre a proposito delle scuole di specializzazione: molti ospedali del Sud, nel corso degli anni, rischiano di non avere specialisti o medici altamente qualificati perché, per come è impostato oggi il sistema delle specializzazioni, gli studenti

Il rischio potenziale cui gli ospedali del Sud e quindi i cittadini del Sud vanno incontro è quello di depauperare di specialisti sia gli ospedali, sia gli utenti, perché i cittadini chiederanno prestazioni agli ospedali del Nord aumentando ancora di più la mobilità sanitaria

prevedendo che si individuino, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, ulteriori modalità attuative per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Relativamente al settore delle farmacie si confermano modifiche importanti, importanti, come la farmacia dei servizi, un presidio sociosanitario che orizzontalizza ulteriormente il rapporto tra sistema sociosanitario e territorio.

del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, rappresenta un ammodernamento ispirato ai principi delle direttive comunitarie e alle proposte di modifica di tali direttive, tra le quali figura la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. La norma che stiamo per approvare riordina l'impianto ordinistico in sanità: un assetto nato, come molti hanno avuto modo di specificare, oltre cento anni fa, inizialmente per la pressione dei medici stessi, spinti da ideali progressisti di tutela della parte meno garantita della categoria e dei diritti dei pazienti. Allora le professioni sanitarie erano poco più di cinque, ora sono poco meno di trenta; prima si parlava di sanità, di cura della malattia o dell'infortunio, ora si parla di diritto alla salute, di primato della prevenzione rispetto alla cura ed alla riabilitazione; prima si parlava di un sistema di protezione sanitaria categoriale, ora si parla di un sistema universale e solidaristico. Per queste valide e nobili motivazioni, già varrebbe la pena approvare questo provvedimento senza tentennamenti.

hanno perso quello spirito che aveva contraddistinto la riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978. Prima effettivamente si parlava di medicina scolastica e gli scolari e i discenti venivano valutati dal punto di vista igienico-sanitario. Prima veramente si parlava di educazione alla salute, perché si facevano i corsi di formazione all'interno delle scuole: i bambini e gli adolescenti venivano informati sulle azioni macro che potevano interessarli e su un determinato tipo di alimentazione cui dovevano sottoporsi. Oggi non si parla più di questi temi; oggi c'è veramente il rischio che la prevenzione, che è il *primum* *movens* dell'educazione alla salute, venga messa da parte e anche su questo dovremo lavorare. Ad oggi la riforma degli ordini nella sanità è stata una vera e propria tela di Penelope, sempre incompiuta, ma ora i tempi sono maturi per il cambiamento. Appare evidente che l'impianto di cui trattasi abbia bisogno di un profondo adeguamento normativo nei contenuti, nelle modalità di partecipazione al voto degli iscritti e di funzionamento interno, nonché nelle sue articolazioni. tener conto della dimensione regionale e dell'eventuale superamento o ridimensionamento di quella provinciale e, soprattutto, di un diverso rapporto con i cittadini, in particolare nella gestione attraverso la mediazione del contenzioso. Avviandomi alla conclusione, signora il provvedimento coglie la centralità e la peculiarità della questione dell'assetto professionale nella Sanità e soprattutto guarda agli operatori e alle operatrici che appartengono alle 11 professioni della salute regolamentate

ma la politica, come è stato detto, è mediazione. Certamente, non si è trattato di un parto facile, però non vi è stata conflittualità all'interno della Commissione e, soprattutto, vi è stata piena autonomia e non c'è stata assolutamente alcuna azione contro professionisti o contro professioni che magari vedranno riconosciuti i loro diritti successivamente (mi riferisco ai fisioterapisti e alle altre professioni).

Ad esempio, gli emendamenti e l'ordine del giorno all'articolo 2 hanno chiesto l'inserimento e l'allargamento a nuovi LEA, limiti che peraltro avevo evidenziato; all'articolo 3 si è chiesta la regolamentazione di nuove professioni sanitarie: dall'agopuntore, all'ingegnere clinico, dal chinesiologo al dottore in scienze motorie, dal massofisioterapista all'odontotecnico e all'ottico optometrista, senza il percorso stabilito dall'articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Perfino la relatrice, che più di tutti ha avuto la possibilità di studiare e analizzare il provvedimento, ha avuto la necessità di inserire all'ultimo momento la norma sulle professioni di chimico e fisico. La richiesta di disciplinare alcune professioni sanitarie non ha fatto altro che dimostrare la superficialità del provvedimento, anche perché quegli emendamenti sono stati presentati da stimati colleghi della Commissione sanità, che hanno avuto modo di studiare il provvedimento per due anni, accorgendosi solo all'ultimo minuto di doverlo cambiare, dopo aver votato favorevolmente in Commissione.

non solo non ammoderna il sistema ordinistico delle professioni sanitarie ma, al contrario, ne rafforza la natura corporativa, mantenendo assolutamente inalterate strutture arcaiche e meccanismi poco trasparenti e affatto rappresentativi. È evidente che *in primis* si pone una riflessione generale sull'opportunità che continuino ad esistere ordini professionali, ben potendo le medesime funzioni essere ricoperte e soddisfatte dai Ministeri vigilanti. In ogni caso è chiaro che l'esistenza di tali ordini nella veste di enti pubblici non economici, con connesso potere impositivo paratributario, normativo, regolamentare, disciplinare e consultivo, mal si concilia con la loro volontà di agire al di fuori di ogni regola pubblica ed in piena e totale autonomia. Appare opportuno che tali enti si adeguino a tutte le norme sulla trasparenza e l'anticorruzione, il pubblico impiego, il codice dei contratti, la contabilità pubblica e quant'altro, e che risolvano tutti i conflitti d'interesse che li riguardano. Appare necessario che sia garantito un controllo esterno da parte del Governo, del Ministero vigilante e della Corte dei conti (sia gestionale che giurisdizionale), tenuto conto del notevole patrimonio economico e finanziario che questo sistema gestisce e controlla, sia direttamente che indirettamente (contributi, formazione, immobili, investimenti, fondazioni, casse di previdenza). Alcuni studi hanno rilevato che il sistema economico riferibile agli ordini professionali (incluso l'indotto) corrisponde a circa il 15 per cento del PIL. Il patrimonio immobiliare e mobiliare riferibile agli ordini professionali e alle casse di previdenza è quantificabile in svariati miliardi di euro. Appare opportuno che siano costituiti esclusivamente ordini nazionali in cui confluiscano diverse professioni sanitarie, o al massimo regionali e interregionali, così da garantire servizi amministrativi efficienti per l'utenza e per i medesimi professionisti. Appare altresì Appare altresì necessario eliminare tutti quei conflitti d'interesse (ad esempio, tra ordini e formazione) che minano il libero sviluppo ed esercizio delle professioni. Sono già entrato nel merito delle incongruenze dell'istituzione delle due professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico, peraltro con due percorsi diversi, per cui non entro nello specifico, ribadendo comunque, in questa fase, che abbiamo valutato il metodo e non la sostanza. Interessante anche notare che compare un articolo (articolo 13) sulla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, che va ad inquadrare il personale nelle rispettive qualifiche, collocandolo in un unico livello. Ovviamente, la rimodulazione avviene aumentando lo stipendio, che viene compensato dalla riduzione del personale per pensionamenti (circa due, tre all'anno), visto che il *turnover* è fissato al 20 Molto interessanti sono le motivazioni che sottendono questo articolo, ovvero il divario economico tra personale del Servizio sanitario nazionale, cui compete una indennità di esclusività del rapporto di significativa consistenza economica e l'omologo personale del Dicastero, cui non è riconosciuto siffatto emolumento. La relazione tecnica ci dice che «La disposizione non impatta significativamente sulla regolare programmazione». I calcoli sono stati fatti sul personale al 31 dicembre 2013, forse, dopo tre anni, sarebbe opportuno verificarli, vedere se la organizzazione funzionale del Ministero è ancora valida e se tutti i dirigenti meritano davvero la nuova qualifica. Forse vi siete dimenticati della meritocrazia. Anche l'articolo 10, contenente disposizioni in materia di formazione medica specialistica, lascia qualche perplessità. Esso consente l'inserimento dei medici in formazione all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa. Praticamente lo specializzando, come ha già sottolineato qualche collega in precedenza, negli ultimi anni della specializzazione, viene inserito «anche per ciò che attiene alla graduale assunzione di compiti assistenziali e all'esecuzione di interventi» nell'attività nell'attività routinaria assistenziale, percependo come stipendio, l'assegno riferibile alla borsa di studio. Praticamente si utilizza un medico, pagandolo meno, ma affidandogli gli stessi compiti di uno strutturato, vicariandone la presenza. Avremo che le strutture sanitarie faranno a gara per avere medici in formazione, che lavoreranno più degli strutturati, perché devono imparare, ma pagati la metà. Non so se vi rendete conto, ma state regolamentando lo sfruttamento dei giovani medici. Per questa e per altre ragioni, che il tempo a disposizione non mi consente di esplicitare, il Movimento 5 Stelle voterà contro questo provvedimento. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario,

ma credo di buonsenso e condiviso da tutti: l'individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici. Mi auguro veramente che il Governo semplifichi la loro in modo da ridurre i lunghi tempi di attesa e di risposta da parte dei comitati etici, soprattutto quelli regionali, perché penalizzano nel nostro Paese, rispetto agli altri Paesi europei, gli operatori del comparto. Un secondo punto fondamentale dell'articolo 1 è, per me, lo specifico riferimento alla medicina di genere. Il tema è stato proposto da questo ramo del Parlamento sin dal 2003, con mozioni ai Governi per sensibilizzare il loro intervento a questo proposito. Ricordo a tutti i colleghi che la medicina di genere, branca innovativa della ricerca biomedica, offre nuove prospettive per il futuro della salute. Sin dal 1992 il Dipartimento della salute americano costituì un ufficio sulla salute della donna; nel 2002 l'OMS costituì il Dipartimento per il genere e la salute della donna; nel 2005 è nato il Progetto salute donna presso il Ministero della salute e abbiamo *master* universitari e cattedre - come, ad esempio, a Padova - di Medicina di genere. Non posso quindi che rallegrarmi con il Ministro per questo passo avanti. Per quello che riguarda l'articolo 2, sembra che finalmente si aggiornino i LEA, garantendo, oltretutto, di partorire in sicurezza con il controllo del dolore nella fase travaglio-parto con tecniche di anestesia loco-regionale, sempre su scelta della paziente. Questo era già stata inserita nei LEA dal ministro Turco anni fa, ma a iso-risorse, cioè senza finanziamenti e quindi demandando il problema alle Regioni, con una diffusione del diritto riconosciuto sempre a macchia di leopardo, con dati incerti e servizi organizzati in modo diverso da una Regione all'altra. Arriviamo ora all'articolo 3 e al riordino delle professioni sanitarie. Credo che in Commissione si sia raggiunto un buon punto di equilibrio, con un ampissimo dibattito e 36 audizioni. Si ridisegnano ruoli e si ridà dignità professionale a più di un milione di operatori che aspettano questo provvedimento, come già ricordato più volte, da più di venti anni.

n. 573 del 2011 che però, come è stato ricordato, non poté andare oltre per motivi politici. Vorrei ricordare un aspetto che ritengo importante: le professioni sanitarie devono essere fuori da un ragionamento di liberalizzazione generale, perché hanno il compito fondamentale di proteggere i cittadini dall'abusivismo, facendo in modo che possano rivolgersi a professionisti laureati con esami di laurea automaticamente abilitanti, a differenza, ad esempio, di altri ordini, come gli avvocati che devono dare un esame per l'abilitazione. A questo proposito, visto che si è a lungo discusso sul riconoscimento della professione di osteopata, anche per le critiche che ci sono piovute addosso, vorrei ricordare, come giustamente ha sottolineato la relatrice, la presidente De Biasi, che non si fanno leggi contro qualcuno o per Si danno infatti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, sì da potersi iscrivere all'albo presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione. Importante è l'ordinamento delle professioni sanitarie di biologo e psicologo. Importante è l'articolo 6, che istituisce l'elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici presso l'Ordine degli ingegneri. Questo è il giusto riconoscimento di una figura professionale a cavallo tra l'ingegneria, la sanità e la medicina, il riconoscimento della scelta effettuata da 4.000 studenti che, dal 2007 al 2015, sono diventati ingegneri clinici

la sicurezza per i pazienti e gli operatori nell'utilizzo appropriato dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche, con compiti di collaudo, manutenzione e gestione operativa, oltre alla gestione del rischio. Importanti sono le relative sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. Estremamente condivisibile è l'articolo 9 con l'aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o sociosanitarie, residenziali o semiresidenziali. Come molto importante è aver messo nero su bianco i criteri per la formazione e anche con l'istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute norme di accesso regolamentate. In conclusione, siamo sulla buona strada. Mi auguro che la Camera esamini velocemente il testo da noi licenziato e annuncio il voto favorevole di Forza Italia.

e colleghi, vorrei anche io unirmi alle parole di coloro che, prima di me, hanno ringraziato innanzitutto la relatrice, senatrice De Biasi, per la tenacia, la pazienza e la determinazione con la quale in questi due anni ha guidato la Commissione

con la voce del collega, senatore Gaetti, abbia espresso delle perplessità che mai, in questi due anni, sono state espresse in occasione del dibattito in Commissione. Forse, così come su alcuni punti abbiamo lavorato intensamente, potevamo lavorare intensamente anche sugli aspetti che oggi sono stati sollevati. Ma capisco che possano esserci altri argomenti che portano ad assumere una posizione contraria, ancorché all'interno della Commissione sanità i provvedimenti siano stati approvati, nella grandissima maggioranza, all'unanimità dei componenti della Commissione.

e le riorganizzazioni che in questo momento in tutte le Regioni sono in atto, con senso di responsabilità e con dedizione. Credo sia ingeneroso qualificarli statali, perché non lo sono, trattandosi di operatori pubblici e privati, e poi perché forse sarebbe bene che cominciassimo a evitare di denigrare i dipendenti pubblici in modo generalizzato e che fossimo più intelligentemente attenti alle luci e anche alle ombre che i molti dipendenti pubblici hanno nel momento in cui svolgono la loro funzione.

consente di fare una manutenzione legislativa e apportare un aggiornamento e un ammodernamento a una disciplina che, in alcuni ambiti, come abbiamo sentito dire più volte, risale al 1946,

per garantire che anche nel nostro Paese le sperimentazioni cliniche si adeguino agli *standard* internazionali (soprattutto quelli dell'etica, della trasparenza e dell'indipendenza dei ricercatori) e che si sappiano governare i conflitti di interesse che in questi settori molto spesso si verificano. Ci auguriamo che il Governo adotti rapidamente i decreti legislativi attuativi di questa che è l'unica delega che viene data al Governo.

produce dei miglioramenti alla normativa esistente che, apparentemente, possono sembrare lontani dagli interessi dei cittadini, ma che in realtà possono avere degli effetti sulla salute delle persone e sui diritti dei cittadini, che cercherò di approfondire rapidamente, nel tempo che mi è consentito. Mi riferisco, in particolare, alla disciplina degli ordini professionali, disciplina degli ordini professionali, che probabilmente - a mio giudizio erroneamente - può essere giudicata da molti una questione tutta interna al mondo delle professioni. Anzi, qualcuno potrà pensare che sia addirittura interna principalmente al mondo dei medici

in questa sede. Se fosse così, non avremmo reso un buon servizio al Paese. In realtà non è così, perché la disciplina che rivede la normativa in tema di ordini professionali ha, in primo luogo, l'obiettivo di dare garanzia ai cittadini. Inoltre, nonostante la lunga storia degli ordini contenga al proprio interno episodi in cui il bene del paziente non sempre è stato messo al primo posto, voglio sottolineare quanto questo riordino in corso di approvazione possa, al contrario, costituire un passo importante proprio proprio nella direzione di fissare delle regole a tutela del paziente. Infatti, assegniamo a tutti gli ordini una nuova missione che è quella di promuovere l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità nell'esercizio delle professioni sanitarie e di valorizzarne la funzione sociale

riconoscendo gli ordini non soltanto alle professioni che tradizionalmente erano costituite in ordini ma anche a tutte quelle professioni di cui abbiamo parlato lungamente in occasione del dibattito, alle alle quali riconosciamo un valore importante nella garanzia dell'assistenza ai cittadini che hanno bisogno di essere tutelati quando perdono la loro salute. Questo provvedimento pertanto aiuta anche a superare in parte quel muro di resistenze che molto spesso c'è nel favorire

Ho sentito dire in molte occasioni, nel dibattito di oggi, che si poteva fare di più. Certo, si può sempre fare di più. Peraltro, un provvedimento che arriva dopo settant' anni si deve dare delle priorità perché può fare quello che è possibile fare quello che è possibile fare alla luce del contesto complessivo e delle condizioni esistenti. Voglio qui ricordare, ad esempio, una richiesta che pressantemente in queste ultime settimane ci è arrivata da parte dei laureati delle scienze motorie. motorie. Nessuno non riconosce il valore che ha l'attività fisica nel promuovere la salute dei cittadini e nell'evitare le complicanze che in qualche caso, in alcuni pazienti, possono verificarsi, ma ovviamente la loro richiesta esula dal confine di questo provvedimento, quindi non può che essere presa in considerazione, eventualmente, in un qualche futuro momento in cui ci sarà una riflessione su questa e su altre professioni. Ricordo, infine, l'articolo 9, che introduce per la prima volta le circostanze aggravanti per i reati contro la persona quando il fatto in danno della persona è commesso nei confronti di persone ricoverate in ospedale

alla fine riuscirà a vedere la luce, almeno in questa Camera. Ci auguriamo che la Camera dei deputati riuscirà a breve a completare l'*iter*, in modo che possa essere definitivamente applicato. un recente articolo di Michele Ainis, le norme e i diritti delle persone vivono solo se c'è un popolo che vi si affeziona, che li sa coltivare, che li assume come guida nei comportamenti quotidiani. Qui abbiamo bisogno che queste norme siano assunte nei comportamenti quotidiani degli operatori e dei responsabili delle politiche per la salute

e alle tante istituzioni che hanno il dovere di farla vivere e di farla applicare: il Ministero della salute, il Ministero della pubblica istruzione, le Regioni, gli ordini professionali e tutti i professionisti del settore sanitario. Un piccolo pezzo a miglior tutela della salute dei cittadini oggi può essere approvato dal Senato. Per questa ragione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento che stiamo per approvare.

nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***

la qualità e anche la cortesia con cui ha seguito il provvedimento

da varie forze politiche, la cui genesi risale alla scorsa legislatura, con una proposta di iniziativa dell'onorevole Livia Turco.

Colleghi, se voi urlate in questo modo, io vado avanti a scampanellare. Consentite alla relatrice di parlare senza essere interrotta. *(Applausi La norma non é stata pensata soltanto nelle Aule parlamentari, quanto piuttosto è nata in gran parte da esperienze già presenti nella società ad iniziativa del terzo settore, di associazioni di famiglie, di fondazioni e di enti locali. Essa testimonia dunque la bellezza del legiferare, quando si intercettano i bisogni delle persone, della società in cambiamento, delle comunità locali e quando il legislatore interviene a dare una cornice giuridica ad un cammino già intrapreso nei territori, accompagnando e sostenendo un modello di *welfare* locale, fatto di sperimentazioni che mettono in gioco competenze, professionalità, sussidiarietà orizzontale e collaborazione proficua tra pubblico e privato. Quindi trattiamo di una normativa una normativa molto attesa da anni e per la quale, per la prima volta, con questo Governo, si prevede già uno stanziamento di risorse nella legge di stabilità, nella quale è stato istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni di euro per il 2017 e di 56,1 milioni di euro per il 2018. Si é discusso anche in queste Aule sull'adeguatezza delle risorse, ma a questo proposito occorre sottolineare due aspetti, entrambi richiamati dalla norma. Il primo riguarda l'importanza dell'istituzione di un Fondo specifico nazionale per una materia in gran parte di competenza regionale, Fondo che diventa però, come richiamato dall'articolo 4 del provvedimento, un un contenitore che è possibile alimentare con la compartecipazione, delle Regioni, degli enti locali, degli enti del terzo settore, di famiglie che si associano, di soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore e che, per le attività di programmazione, prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. Il secondo aspetto, a proposito di risorse, ma che riguarda anche il rapporto di questa normativa con tutta l'impalcatura legislativa già esistente, sia nazionale che regionale, viene chiarito e specificato meglio nel testo della 11a Commissione rispetto a quello Camera. In sostanza, a premessa dell'articolo 2, si collega il provvedimento in esame con il quadro normativo già esistente. È un provvedimento, inoltre, con una platea definita: le persone con disabilità grave, secondo quanto prevede l'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come è disciplinato nella finalità della legge. Il legislatore interviene dunque prendendosi cura delle maggiori fragilità presenti tra i nostri cittadini e le nostre cittadine e delle loro famiglie. Abbiamo realizzato, in Commissione lavoro, audizioni importanti con associazioni, professionisti e organizzazioni di rappresentanza, ed in questo periodo ho avuto modo di visitare molte strutture, incoraggiare in qualche Comune esperienze innovative di residenzialità, come la costituzione di gruppi appartamento per persone con disabilità, e di incontrare molti genitori. Qualche settimana fa, in un incontro pubblico, un padre, prendendo la parola, ha sottolineato: «parlo io, perché mia figlia non può». Sappiamo che la normativa ricomprende in gran parte persone con disabilità intellettiva, dunque il disegno di legge si rivolge a chi, molto spesso, non può esprimere i propri desideri, a chi non può far valere i propri diritti. Ebbene, colleghi e colleghe, il Parlamento italiano, votando questo disegno di legge, darà voce a chi spesso voce non ha e rassicurerà tanti genitori sulla sorte dei propri figlioli quando non potranno più essere loro vicini. La legge riprende la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall'Italia nel 2009, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e a sostenere una vita autonoma con l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità. È una legge che si propone di intercettare bisogni di grande umanità, la serenità delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La serenità si assicura innanzitutto progettando un percorso di vita, il durante e il "dopo di noi". Questo collegamento è stato richiesto dalla gran parte dei genitori, delle famiglie e da tutti i soggetti auditi in Commissione. Sono proprio questi bisogni che hanno guidato la nostra attività di miglioramento, in Commissione lavoro, del testo pervenuto dalla Camera. I genitori delle persone con disabilità sono messi nelle condizioni, con questo provvedimento, di guardare al futuro partendo dal presente, dalle situazioni che vivono quotidianamente. Infatti, la normativa, al comma 2 dell'articolo 1, riprende quanto già stabilito da una delle leggi più belle e importanti della storia legislativa italiana, la legge n. 328 del 2000, purtroppo in gran parte inattuata. L'articolo 14 della suddetta legge stabilisce la predisposizione di un progetto individuale per le persone con disabilità. Dopo l'approvazione di questo disegno di legge, con il miglioramento apportato in Senato, il progetto individuale deve essere integrato con le misure previste da questo disegno di legge, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Nelle finalità della legge, in Commissione abbiamo inoltre rafforzato la soggettività delle persone con disabilità e il ruolo di sostegno dei genitori, per evitare che si lasciasse erroneamente intendere che questi ultimi fossero gli unici responsabili dell'assistenza. Sempre per andare incontro alle esigenze dei genitori, delle famiglie, all'articolo 1, comma 3, durante i lavori della Commissione, ho raccolto da relatrice le istanze di tutti i soggetti auditi e di gran parte delle proposte emendative dei colleghi di maggioranza e di opposizione, al fine di dare la possibilità alle famiglie, per poter usufruire di agevolazioni fiscali, di scegliere a chi assegnare e come proteggere il patrimonio da destinare all'assistenza, la cura e la protezione dei propri figli. disegno di legge, così come approvato in prima lettura, prevedeva la possibilità, per le famiglie con persone con disabilità, di poter utilizzare il solo *trust* come strumento di tutela del patrimonio dopo la morte dei genitori. La norma oggi è stata migliorata, offrendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche istituti già previsti dal nostro sistema normativo, in particolare dal codice civile. Per questa ragione è stata introdotta la possibilità di segregare e tutelare il patrimonio a favore delle persone con disabilità utilizzando l'articolo 2645-*ter* nonché i fondi costituiti per mezzo di contratti di affidamento fiduciario assoggettati a vincolo di destinazione anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel settore della beneficenza. Per quest'ultima possibilità offerta dalla norma si valorizzano le esperienze già esistenti di solidarietà e sussidiarietà da parte di organizzazioni filantropiche. In questo modo viene data l'opportunità ai familiari di ottenere la segregazione del patrimonio ovvero la tutela dello stesso per tutta la durata della vita della persona con disabilità, proteggendolo da eventuali azioni da parte dei creditori, perché questo va incontro alle maggiori preoccupazioni dei genitori. Peraltro, la previsione di diversi istituti fruibili da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla tutela, anche dopo la morte, delle persone con disabilità, risponde alla volontà di favorire il più possibile l'adozione di forme di cura e di assistenza, consentendo la scelta dello strumento che meglio si adatta alle differenti esigenze delle famiglie. In coerenza con quanto sopra, sono state introdotte specifiche disposizioni, finalizzate ad evitare utilizzi strumentali sotto il profilo fiscale o comunque non in linea con le finalità La modifica al comma 3 dell'articolo 1, naturalmente va a riscrivere l'articolo 6. Per gli istituti di tutela patrimoniale, la norma prevede che siano esenti dall'imposta di successione e donazione; l'esenzione permette ai genitori, o anche ai soggetti terzi interessati alla tutela delle persone con disabilità, di trasferire il patrimonio da destinare senza alcun aggravio di imposta. In questo modo, si intende favorire - questa è la bontà della legge - l'utilizzo degli strumenti a tutela della persona con disabilità, evitando che il pagamento dei tributi possa ridurre in modo considerevole le risorse da destinare allo scopo che si prefigge il disegno di legge. Il comma 2, specifica che l'esenzione e l'agevolazione di cui all'articolo 6 perseguono come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza. Naturalmente, questa modifica allarga agli altri

I commi 4 e 5, invece, rappresentano un novità rispetto al testo della Camera. Il comma 4, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni, nonché l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, quando, a seguito della premorienza del disabile rispetto ai soggetti che hanno istituito il *trust* o stipulato fondi speciali e tutti gli altri istituti previsti, i beni e i diritti vengano trasferiti a favore di questi ultimi. Si intende tutelare in questo modo i familiari della persona con disabilità in caso di premorienza di quest'ultimo, evitando che la retrocessione dei beni possa subire un prelievo fiscale che contrasterebbe palesemente con le finalità della norma. Il comma 5, prevede che il trasferimento del patrimonio residuo - sul patrimonio residuo ci sono state molte richieste da parte dei soggetti interessati - sia soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, che dovrà essere applicata tenendo presente il rapporto di parentela intercorrente tra disponenti, fiducianti e destinatari del suddetto patrimonio. Questa precisazione si è resa necessaria per evitare che, al momento di scioglimento del *trust* o della cessazione del contratto di affidamento fiduciario, possano essere realizzate successioni in esenzione di imposta, ogni qual volta tra i soggetti beneficiari sia presente un soggetto disabile. In sostanza, una volta venuto meno il bisogno di assistenza della persona con disabilità, sarà possibile trasferire a terzi il patrimonio, assoggettandolo a tassazione secondo i criteri ordinari.

Il Governo, con un decreto apposito, dovrà definire, insieme alla Conferenza Stato-Regioni, gli obiettivi di servizio ed entro sei mesi si dovranno definire i criteri di accesso.

Una volta approvata, questa legge sul "dopo di noi" deve richiedere uno sforzo di responsabilità da parte della classe dirigente nazionale e regionale per colmare una lacuna, ormai non più tollerabile, di attuazione delle normative attuali, per garantire l'esigibilità dei diritti su tutto il territorio nazionale alle persone con disabilità. L'articolo 4, fornisce indirizzi in tema di destinazione del Fondo nazionale, avendo sempre fermo l'obiettivo di tendere alla deistituzionalizzazione, come stabilito nelle finalità della legge e andando a finanziare esperienze innovative di residenzialità, come *co-housing* e gruppi appartamento. Mi sta a cuore sottolineare una precisazione sullo spirito della norma, come definito dal testo approvato dalla Camera, sul punto *b)* dell'articolo 4, perché sono emerse delle preoccupazioni nel corso delle audizioni. Gli interventi temporanei si renderanno necessari solo ed esclusivamente per tamponare situazioni di emergenza che si possano venire a creare per cause impreviste e imprevedibili. quindi adottate misure temporanee, per evitare che le persone con disabilità grave possano trovarsi senza un supporto abitativo.

articolo non è stato modificato dal lavoro della Commissione. Il tema delle polizze assicurative è particolarmente delicato ed importante ed importante per migliorare gli strumenti a disposizione delle famiglie a tutela delle persone con disabilità. È auspicabile che questo tipo di agevolazione possa essere ampliato in futuro, costruendo un percorso di approfondimento legislativo in grado di assicurare un trattamento fiscale agevolato per quelle famiglie che scelgono di tutelare le persone con disabilità disabilità mediante lo strumento della polizza assicurativa. In questo caso si potranno prevedere vincoli specifici all'utilizzo ed alla destinazione delle disponibilità ancorando il regime fiscale agevolato alla effettiva presenza di vincoli contrattuali stringenti volti a favorire il soggetto disabile. Molto importanti sono gli articoli 7 e 8 del provvedimento, in cui si stabiliscono (articolo 7) campagne informative per far conoscere le norme e (articolo 8) le modalità del monitoraggio che il Parlamento dovrà effettuare sullo stato di attuazione della legge.

Abbiamo ereditato questa esigenza, condivisibile, dalle osservazioni che sono emerse dal dibattito alla Camera e in particolare dagli spunti che la relatrice del provvedimento, l'onorevole Carnevali, ha fatto emergere nel corso della relazione in Aula, nonché da richieste emendative avanzate da alcuni colleghe e colleghi in Senato. come ci ha evidenziato in Commissione lavoro il qualificato apporto del presidente dell'ISTAT Giorgio Alleva, dovremmo avere maggiori dati amministrativi per conoscere meglio le persone con disabilità e per meglio legiferare. Conoscere meglio le persone con disabilità grave è un impegno che attraverso questa legge ci prendiamo, per seguirle, attraverso il monitoraggio previsto, perché possano vivere una vita di benessere e autonomia con i loro genitori, ma anche quando i genitori non ci saranno più.

In un incontro pubblico non più tardi di ieri, una madre mi ha detto che queste norme intercettano le fragilità, perché «le fragilità non sono un mondo a parte, ma una parte del mondo». È questo il "dopo di noi".

oserei dire che oggi, come ha detto la relatrice, è un giorno particolarmente importante. Mi rifaccio ai dati statistici dell'ISTAT riferiti agli anni 2012-2013,

89.000 di età superiore ai sessant'anni vivono con genitori anziani, 52.000 persone disabili vivono da sole

aumentare la rete di protezione attraverso regimi fiscali agevolati per l'assistenza ai disabili, di attivare percorsi per l'indipendenza degli individui con disabilità gravi, creare case famiglia, ovvero comunità, ovvero coabitazioni di disabili in appartamenti a ciò dedicati, anche per evitare il ripetersi di casi di segregazione, alcuni dei quali segnalati anche dalle cronache. istituire il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi e prive del sostegno familiare, nonché di elevare il limite delle detrazioni

Al di là del ritardo del *welfare* in Italia, purtroppo occorre segnalare che le ultime leggi di stabilità hanno notevolmente ridotto i trasferimenti finanziari a livello locale (quindi ai Comuni) per il settore sociale.

A copertura degli oneri della legge vengono utilizzati i 90 milioni appostati in un fondo presso il Ministero del lavoro per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno famigliare, tale somma non copre minimamente la riduzione dei trasferimenti operati a carico degli enti territoriali. Peraltro, il Patto di stabilità impedisce ai Comuni di mettere in atto alcune misure per il sociale inoltre che i tempi per l'applicazione e l'emanazione dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal comma 2, articolo 2, del provvedimento in esame

buon lavoro alla relatrice.

al nostro esame si muove nella direzione della tutela del diritto all'autonomia e alla vita indipendente delle persone con disabilità, favorendo il loro benessere e la piena inclusione sociale. Ed invero, è necessario garantire che il cittadino disabile, anche e soprattutto al momento della perdita dell'adeguato sostegno genitoriale, non venga abbandonato dalla comunità. La perdita del sostegno genitoriale è un momento fortemente drammatico per un disabile, per ovvie ragioni. Come noto, vi sono moltissimi casi dove la disabilità di alcune persone è talmente grave da non consentire di svolgere in maniera autonoma nessuna attività legata tanto al proprio essere quanto alle relazioni con il prossimo. disabilità viene comunemente intesa come sinonimo di menomazione, cioè un fatto accidentale che afferisce al fisico, alla mente, ai sensi; è una distanza più o meno grave dalla media della normalità, valutabile, sbrigativamente, con logiche sanitarie. Essa riguarda e risiede esclusivamente nella persona che ne è affetta. Con una maggiore consapevolezza, invece, ci si rende conto di come la disabilità non sia un concetto perpetuo ed inesauribile che possa essere fotografato con un'immagine che non ha scadenza. Essendo il risultato di un'interazione, e potendo modificarsi uno degli elementi di tale scambio, la disabilità che conosciamo oggi potrebbe essere molto diversa da quella di domani (peculiarità diverse, nuove forme di esclusione, nuove forme di partecipazione). Assume, quindi, la forma del paradigma, cioè del modello interpretativo della realtà. La connotazione di gravità viene assunta dall'handicap quando sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sia nella sfera individuale, che in quella di relazione. per tali soggetti la vita non può assumere lo stesso significato che ha per le persone cosiddette normali, e non può neanche definirsi tale. L'attesa di vita ridotta nonché la pessima qualità della medesima non ricade solo sui soggetti affetti da disabilità grave, ma coinvolge le loro famiglie ovvero la loro unica e vera risorsa dal momento che i servizi pubblici in questo settore risentono di note carenze. Pertanto, i valori e i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità devono rappresentare un sistema di riferimento etico anche per il compimento delle scelte future rispetto alla perdita del sostegno genitoriale ossia nel momento del "dopo di noi". Al riguardo, però, occorre effettuare una prima precisazione. Il disegno dì legge in esame dichiaratamente disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone affette da grave disabilita prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi ì genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. sempre che non se ne fornisca un'interpretazione estensiva in tal senso, venga modificato indicando non solamente entrambi i genitori, ma anche chi ne fa le veci esercitando la responsabilità genitoriale. Il benessere del disabile deve essere oggetto di costante monitoraggio attraverso la definizione, con continua implementazione, di progetti di vita che non possono di certo assumere le caratteristiche delle sperimentazioni. La persona con disabilità va presa in carico e seguita nell'arco della vita, assecondando le sue inclinazioni e potenzialità e supportandola insieme alla famiglia verso l'autonomia. Ciò è possibile solo se si uniscono le competenze, si integrano le risorse e le si assicurano per tutto l'arco dell'esistenza. Così come si rende imprescindibile una valutazione di impatto ed un costante monitoraggio degli effetti delle varie politiche sociali che seguiranno l'emanazione di tale Pertanto, diversi elementi del testo di legge andrebbero rafforzati ed altri definiti con maggior dettaglio, attraverso una loro modulazione che tenga conto di alcune delle indicazioni fornite nel ciclo di audizioni svolto in 11a Commissione delle associazioni e ONLUS italiane che operano A titolo esemplificativo, occorrerebbe prescrivere una tempistica tecnica, nel caso particolare dei cittadini disabili privi di sostegno familiare, dei livelli essenziali di prestazioni nel campo sociale (che si immagina congrua in un termine non superiore a centoventi giorni). Inoltre, si chiede una coerenza di fondo nella filosofia che ispira il presente disegno di legge: è possibile prendersi cura delle persone con disabilità nella propria dimora e farlo è una scelta giusta; permettere a chi è in gravi difficoltà di vivere la propria esistenza con dignità significa realizzare quanto la Costituzione prescrive. Pertanto, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale suddetti devono essere garantiti privilegiando (ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328) i servizi di aiuto e di sostegno per favorire la permanenza a domicilio, le strutture semiresidenziali e i centri di assistenza e accoglienza a ciclo diurno. Occorre infatti avere come priorità la deistituzionalizzazione e la domiciliarità, rafforzandole attraverso una loro maggiore esplicazione nel testo di legge al nostro Infatti, anche se indicate come obiettivi, esse potrebbero finire per non essere preferite ad altre misure semmai già rientranti nelle attuali "previsioni residenziali", restando, in tal modo, lettera morta. Sul punto, occorre formulare qualche osservazione in merito all'articolo 3 del disegno di legge laddove lo stesso subordina l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale norma potrebbe essere ampliata attraverso la previsione che il decreto suddetto stabilisca che le misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo debbano essere adottate prioritariamente per attivare processi di deistituzionalizzazione per il rientro

dei singoli beneficiari. Del resto, in tal senso va l'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il quale prevede che gli Stati assicurino ad esse l'accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione.

che il Fondo previsto, ma anche tutte le politiche messe in atto per la disabilità, possano contribuire a riprodurre strutture in contrasto con i principi propri della Convenzione ONU. Occorre, pertanto, ribadire la necessità di un'effettiva integrazione sociosanitaria attraverso la quale le ASL e gli enti locali, in collaborazione con cooperative sociali, fondazioni e associazioni di famiglie, possano affrontare il tema del durante e del "dopo di noi". Occorre, al contempo, stabilire le modalità per la verifica dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni domiciliari, residenziali e semiresidenziali. Pertanto, ritengo utile cogliere questa ultima lettura per rafforzare un disegno di legge ancora troppo

*(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, in questi giorni il Parlamento e l'opinione pubblica finalmente sono stati fortemente impegnati nel dibattito sui diritti civili e la politica si sta occupando del cambiamento della società e della sua cultura. È bene che anche su altri temi si ragioni sempre a partire dalla fotografia della realtà dando alle indagini statistiche e agli studi sui cambiamenti sociali, condotti il più delle volte a prescindere dalle scelte politiche, la giusta centralità. Il provvedimento, finalmente all'esame definitivo, è frutto della consapevolezza che attualmente c'è uno Stato sociale italiano che va modificato tenendo conto di esigenze particolari di cura e benessere molto diverse rispetto a qualche decennio fa. Poco se n'è fatto negli anni addietro. I mutamenti sociali e demografici hanno stravolto i rapporti di cura che legavano, in un circuito virtuoso di reciproca assistenza, nonni, figli e nipoti. Se questo vale per tutte le famiglie, ancor più riguarda le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità gravi, per le quali, oltre alla fatica quotidiana, si aggiunge l'angoscia per il futuro nel momento in cui coloro che danno cure e assistenza non ci saranno più. Questa proposta di legge nasce dalla volontà di dare una risposta a questa angoscia e spostare le preoccupazioni del "dopo" dalla famiglia all'intero contesto sociale. Noi vogliamo dare alle famiglie e alle persone con disabilità la possibilità di progettare il proprio futuro, mettendo a disposizione strumenti e risorse che non vogliono certo imporre un percorso *standard* - altrimenti che libertà di scelta ci potrebbe essere ma tanti possibili percorsi tra cui scegliere quello più rispondente alle esigenze e alle preferenze della famiglia. Questa legge dà la possibilità di uscire dalla logica di progetti finanziati per un lasso limitato di tempo, per concentrarsi su progetti di vita a lungo termine; non è semplice per i familiari affrontare e sostenere il percorso di crescita di un figlio disabile; spesso si ha paura di affidarlo a strutture idonee producendo solitudine e isolamento sia ai disabili, che alla famiglia. Uno degli scopi del provvedimento in discussione, è proiettare le famiglie nella giusta direzione e serenità mentale, sapendo che ci sono persone che si occuperanno dei propri cari disabili in modo ottimale. Una delle preoccupazioni più forti per i genitori di persone disabili riguarda il dopo, il momento in cui essi diventeranno anziani e non potranno più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana e soprattutto il momento in cui i genitori non ci saranno più il figlio disabile dovrà trovare chi lo assiste. Sono convinta che oggi stiamo facendo un passo civile importantissimo: stiamo dando la possibilità di vivere al meglio e di dare una qualità e una risposta dignitosa alla vita di questi ragazzi e di Stiamo dando precisi diritti a persone che non sono autonome e alle quali è venuta meno la rete del supporto familiare, il diritto a veder rispettato il proprio diritto alla vita e alle cure necessarie, che esige risposte concrete e che rappresenta un dovere a tutti i diversi livelli istituzionali. Il mondo della disabilità ha progressivamente vissuto profonde trasformazioni. Da diversi anni c'è stata un'azione di rinnovamento dei servizi e degli interventi a favore del disabile. Ma il vero cambiamento si è avuto con una vera e propria integrazione e non più una semplice inclusione sociale per le persone disabili; quindi un processo più complesso che ha visto il coinvolgimento dell'intero tessuto sociale, un processo di cooperazione e di coordinamento di tutti, istituzioni e non. Una parte importante è stata fatta dai disabili stessi, assicurandosi una partecipazione lavorativa; quindi produzione, realizzazione e competitività con il resto del mondo, coniando l'espressione «diversamente abili» per la maggior parte di loro rimane l'esigenza principale e vitale di assicurarsi un servizio di assistenza che renda meno gravosa l'insostenibile pesantezza del quotidiano per i loro familiari, specialmente per quelli con handicap gravi o con esigenze particolari. Ed ecco l'intervento cruciale e mirato del Parlamento in sintonia con il Governo, con la legge che stiamo per approvare. Si tratta di aiutare ad attivare un processo graduale che prende in considerazione vari aspetti: economici, sociali, organizzativi. Un passaggio graduale che va fatto "durante noi", dagli aspetti relazionali ed affettivi a quelli più concreti, positivi e reali. Ringrazio tutti i colleghi della Commissione lavoro per il sostegno e il lavoro svolto in questo provvedimento. In modo particolare ringrazio la relatrice, senatrice Annamaria Parente, per

La modifica più rilevante apportata in Commissione riguarda l'articolo 6, finalizzata ad ampliare, oltre al *trust* previsto dal disegno di legge arrivato dalla Camera, la tipologia di strumenti utilizzabili dalle famiglie per conferire beni e diritti ai propri figli. Si prevedono anche vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come poc'anzi detto dalla relatrice. Mi avvio alla conclusione. Il secondo emendamento approvato riguarda l'articolo 1 e va a rafforzare l'idea del progetto per l'autosufficienza della persona con disabilità, prevedendo un maggior rispetto delle sue volontà, ove è possibile, e di quelle dei genitori o di chi ne tutela gli interessi.

il disegno di legge che ci apprestiamo a esaminare oggi in Assemblea reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno.

dei deputati, che in Senato si è assistito a una vera condivisione trasversale e a un interesse da più parti, certamente scaturiti da una decisa volontà politica nell'affrontare questo tema molto delicato, per colmare una volta per tutte un profondo vuoto legislativo - e non solo - che investe la nostra società ormai da troppo tempo. trattato del risultato di un percorso lungo e travagliato, senza che mai si vedesse la luce, dato che per troppo tempo la politica non è riuscita a dare le giuste risposte in maniera concreta e tempestiva, oltre la semplice retorica. Il provvedimento in esame vuole dare un nuovo inizio e una nuova speranza a coloro che già lottano ogni giorno per riuscire a vivere una vita normale.

Migliaia di famiglie italiane vivono nell'angoscia e nella paura di non sapere chi si occuperà dei propri figli affetti da disabilità e quale sarà il loro futuro il giorno in cui non ci saranno più.

proprio futuro. Ciò è quanto di più grave ci possa essere: non è certamente bello essere in completa balia del proprio destino. Migliaia di famiglie si stanno facendo carico interamente, con le proprie forze, dei familiari disabili, sotto tutti i punti di vista, e finora hanno rappresentato per questi ultimi il vero ed unico *welfare*.

Difatti, sul tema della disabilità, in Italia vi è una vera e propria lacuna, dovuta, come detto, ad un forte ritardo e alla mancanza cronica di attenzione ad una riforma del *welfare* che prenda in considerazione la struttura sociale esistente, alle esigenze di cura e benessere che stanno mutando nel tempo e che richiedono pertanto nuove e più efficaci risposte. Il provvedimento prevede l'istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare affinché possano essere garantiti percorsi personalizzati per i disabili gravi dopo la morte dei genitori. Verranno pertanto stabiliti progetti di vita personalizzati.

Il Fondo avrà una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2016, di 38 milioni per il 2017 e di 56 milioni annui a decorrere dal 2018. Spetterà poi alle Regioni definire i criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte. È da notare quanto il contributo che inizialmente era stato previsto si sia ridotto progressivamente dall'iniziale che si prevedeva lo Stato potesse concedere per finanziare questa legge. Dal 2017 di prevede uno stanziamento inferiore ai 60 milioni di euro annui; se si prende anche in considerazione il fatto che i Comuni italiani spendono circa sette miliardi per la disabilità e 1,5 miliardi per i disabili privi di sostegno familiare, il tutto ci appare davvero ben poca cosa. I trasferimenti erariali ai Comuni per il sociale continuano a vedere una diminuzione e molto spesso gli stessi Comuni sono costretti a subire queste riduzioni proprio per i vincoli di bilancio del Patto di stabilità portati avanti da questo Governo, che comprimono ogni manovra utile al riguardo. Noi come Gruppo di Forza Italia, interessati da sempre alla politica a difesa della famiglia e dei suoi individui, valutiamo con favore iniziative che vanno a tutela di un patrimonio così sacro per la nostra società. Il provvedimento in questione può rappresentare davvero un segnale di speranza per tutte quelle famiglie che si trovano a vivere tale situazione, che si potranno sentire non più sole avranno la giusta e dovuta attenzione da parte della politica. Ne va certamente del futuro di queste famiglie, ne va del futuro di queste persone che sono meritevoli come tutti noi altri di poter vivere una vita dignitosa e serena. È diritto di queste famiglie poter vivere senza il terrore per il futuro dei propri figli.

presentato in 7a Commissione, riguardante un fatto di attualità molto increscioso che sta accedendo in questi giorni e, purtroppo, già il 1° 1° giugno ci sarà un'udienza della giustizia sportiva al riguardo. Mi riferisco al caso clamoroso della Virtus Lanciano, squadra di serie B abruzzese, che in questi giorni sta subendo un trattamento dalla giustizia sportiva assai poco equiparabile a quanto accaduto in tante altre vicende simili. Chiedo, quindi, con la massima urgenza, che mi venga data risposta all'interrogazione perché dev'essere fatta piena luce sulla conclusione del campionato di serie B, che vede, appunto, una squadra abruzzese, la Virtus Lanciano - già giudicata dalla giustizia sportiva con sentenza favorevole di riattribuzione di tre punti fondamentali per la classifica fatta oggetto nuovamente di una ulteriore procedura di giudizio: caso forse unico nella storia del calcio. Si tratta tra l'altro di un provvedimento per ritardato pagamento, mentre per la compravendita di partite, cosa assolutamente indecorosa, su cui proprio in queste ore e in questi giorni stanno emergendo fatti sconcertanti, non si usa né la stessa velocità nel giudizio, né così

Quindi, chiedo alla Presidente di sollecitare il Governo, perché il 1° di giugno ci sarà un' udienza al riguardo.

concernente la determinazione e la ripartizione del nuovo Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa delle aziende sanitarie locali. Si tratta di un tema rilevante, poiché dal passaggio dal precedente sistema al nuovo sistema della retribuzione di risultato non sarebbero dovuti emergere oneri aggiuntivi diretti o indiretti. Viceversa, il risultato di tale operazione interpretativa espone le aziende sanitarie, che hanno in corso delle cause, ad un aggravio di spesa assolutamente ingiustificato e insostenibile, stimato in diversi milioni di euro per ciascuna amministrazione, a decorrere dall'anno di costituzione del nuovo fondo di risultato, con un onere totale, relativo all'intero territorio nazionale, valutabile in centinaia di milioni di euro. Perciò sollecito la risposta all'interrogazione citata, nella speranza che lei, signora Presidente, voglia attivarsi affinché venga data una celere risposta, al fine di impedire che si possa causare, da un lato, un enorme incremento di spesa per le aziende sanitarie, assolutamente incompatibile con le attuali disponibilità di bilancio e, dall'altro, un'erogazione di compensi incentivanti retroattivi di valore abnorme.

considerato l'allora imminente avvio della stagione turistica estiva. Il 21 ottobre successivo ho sollecitato la risposta, conscio che la stagione invernale fosse ormai alle porte, senza ottenere risposta alcuna. Il Veneto, da anni, è sul podio quale prima Regione turistica Pertanto l'interpellanza è volta a comprendere se vi sia l'intenzione di ripristinare celermente il collegamento diretto tra Roma, Belluno e Calalzo di Cadore, in vista della nuova stagione estiva, di instradare verso Vicenza e Rovigo la coppia di Intercity Notte Roma-Bolzano, ma soprattutto di prevedere il prolungamento della corsa di un convoglio ad alta velocità, diretto a Verona e ivi terminante la sua corsa, sino alla città di Vicenza. **Interventi

Questi lavoratori hanno ricevuto una lettura di licenziamento e quindi verranno certamente messi in mobilità, visto che sono in un certo numero. Il grande problema è che purtroppo la normativa attuale in materia di appalti consente, in maniera anche purtroppo troppo vistosa, a determinate aziende di non essere obbligate a riprendersi i lavoratori dal vecchio appalto, a meno che ciò non venga inserito all' interno del capitolato.

un confronto serio sull'argomento), inserire la cosiddetta clausola sociale in tutti gli appalti, soprattutto quando si tratta di aziende così grandi come la Finmeccanica.

appalto. Chiedo quindi un intervento del MISE su questa vicenda, perché non possiamo consentire a questi lavoratori di restare per strada, soprattutto in un momento così drammatico che vive l'Italia, e che vive soprattutto il Sud.